Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 843, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, considerato che l'articolo

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo,

ai registri delle associazioni del volontariato delle varie Regioni italiane, possano essere esentate dal pagamento dell'IMU. Ricordo a tutti i colleghi che quando parliamo delle associazioni operanti nel campo dei diversamente abili, quasi sempre ci riferiamo ad associazioni formate da genitori di ragazzi o di famigliari che hanno difficoltà. Quando si pensa, ad esempio, ad un appartamento relativo al mondo della disabilità si pensa a quelle esperienze di autonomia che i genitori fanno spesso fare ai loro figli,

la rideterminazione della rendita catastale degli impianti di produzione di energia ed insieme l'attribuzione dei relativi proventi. La questione è nata nel corso dell'anno 2005 quando fu introdotta un'innovazione importante, che non è riuscita però a trovare concreta attuazione per effetto di una stratificazione di difficoltà successive che si sono sovrapposte sia in termini di individuazione delle modalità per la rideterminazione della rendita catastale in riferimento al calcolo dell'imposta, sia in termini di

nel 2013, lo Stato ha ricentralizzato questa imposta. L'ordine del giorno impegna il Governo a valutare la possibilità di confermare l'attribuzione agli enti locali, nell'entità definita dall'aliquota base, dell'entrata da IMU. Ho parlato di confermare, perché nel frattempo la norma che recentemente il Parlamento ha approvato in ordine ai debiti della pubblica amministrazione ha introdotto il concetto che in sede di accertamento la relativa tassa,

Con l'ordine del giorno G1.106 abbiamo voluto affrontare una questione che purtroppo non ha trovato spazio tra le disposizioni del provvedimento e nei confronti della quale si rende inderogabile un intervento del Governo, volto a chiarire e rettificare la normativa attualmente vigente così come espressa dal provvedimento in esame. Faccio riferimento alla configurazione dell'abitazione di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Nell'ambito della discussione di questo decreto ho provveduto a presentare un emendamento che non è stato accolto, finalizzato a prevedere la sospensione per l'anno 2013 del versamento della prima rata dell'imposta municipale per la suddetta categoria di immobili, ripristinando quindi quanto disposto originariamente dal decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, che aveva stabilito che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considerava direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Purtroppo questa disparità di trattamento, che a partire dal 1993 sembrava non esserci,

provvedimento che ha introdotto il principio di discrezionalità in materia in capo ai Comuni. Considerando le note criticità finanziarie che condizionano i Comuni italiani, molti ovviamente hanno optato per il riconoscimento dell'unità immobiliare come secondaria, con tutte le conseguenze del caso. Paradossalmente, anche per gli immobili considerati abitazione principale dai Comuni si è creata una sorta di vuoto operativo, non beneficiando della sospensione prevista nel provvedimento in in particolar modo, di alcune criticità burocratiche. In considerazione del progetto di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, che dovrebbe essere avviata nel breve periodo, sarebbe auspicabile che in questa sede venisse confermata la volontà originaria del legislatore, che intendeva equiparare lo *status* delle abitazioni dei cittadini italiani dentro e fuori i confini italiani, subordinandolo esclusivamente a talune condizioni, come quella della non locazione. chiediamo dunque un impegno attraverso un gesto di coerenza normativa, oltre che di tutela dei diritti dei nostri connazionali residenti all'estero, i quali spesso sono proprietari di piccole abitazioni, per lo più lasciti ereditari e luoghi di

una discriminazione non soltanto tra cittadini in Patria e quelli all'estero, ma anche e soprattutto tra quelli residenti all'estero, in virtù del citato principio di discrezionalità. Tale situazione, con i riflessi socioeconomici che comporta, rischia di compromettere il legame tra il cittadino e la Patria, di cui l'immobile è espressione tangibile. in questa prospettiva abbiamo il dovere di esorcizzare tutto ciò. Pertanto, abbiamo voluto chiedere un impegno al Governo, nell'ambito della complessiva riforma della disciplina di imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, a rivedere il principio di discrezionalità dei Comuni, prevedendo il riconoscimento automatico come abitazione principale delle unità immobiliari a destinazione abitativa possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

che abbiamo contestato perché interveniva su fatti di ragioneria che non sono certamente di competenza del Parlamento. Al riguardo, anche in futuro, signor Presidente, dovremo cercare di porre attenzione, perché non si può certamente accettare il fatto che il Governo entri nelle competenze parlamentari attraverso lo strumento della Ragioneria. Possiamo accettare i vincoli di bilancio che ci provengono dall'articolo 81 della Costituzione, ma non altri tipi di vincoli, Abbiamo poi appreso che tutti gli emendamenti sarebbero caduti per favorire l'*iter* di questo intervento legislativo e, quindi, abbiamo trasformato ciò che riteniamo essenziale per l'economia del nostro Paese in ordine del giorno. Mi appello al Governo per l'accoglimento di questo ordine del giorno, perché interviene nel settore dell'edilizia che non è solamente un comparto fondamentale per lo sviluppo e la crescita del nostro prodotto interno lordo,

non possono che essere considerati come altri beni strumentali di altri settori della produzione del nostro Paese. Invitiamo quindi il Governo, nella riforma dell'IMU più volte annunziata, a tener conto di questo settore delicato. Tra l'altro, è una forma di intervento anticiclico: in un momento di depressione di un determinato settore di mercato non si può che investire ulteriormente in quel settore per dargli la giusta spinta per la ripresa. È un settore che deve essere attenzionato, e l'intervento del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà è voluto andare in questa direzione, verso cioè atti concreti per lo sviluppo effettivo del nostro territorio. L'edilizia ha inoltre un vantaggio, riesce a coprire tutto il territorio nazionale, da Pantelleria fino a Trento; un intervento di questo tipo diventa quindi davvero strutturale perché ricopre tutto il territorio nazionale e riesce ad espletare gli effetti benefici della propria azione su tante

illustrare l'ordine del giorno G1.100, mi appello non solo al Governo, ma a tutte le forze politiche presenti nel nostro Senato, perché possano dare il giusto sostegno ad un settore che riteniamo davvero trainante per l'economia del Paese.

una menzione particolare per gli ordini professionali in genere e per i liberi professionisti in assoluto, che - voglio ricordare - rappresentano una parte rilevantissima del nostro mercato del lavoro e più in generale della nostra economia. Ricordo solo che in Italia

Se aggiungiamo a questi i praticanti i dipendenti degli studi professionali, raggiungiamo la quota di quattro milioni di lavoratori. essere riconosciuti all'interno di questo decreto, con uno specifico riconoscimento, assume un significato particolarmente importante, anche in considerazione del fatto che

se questo ci sarà chiesto dai relatori, ritireremo l'emendamento 4.20 trasformandolo in ordine del giorno. Chiediamo però che il Governo su questi punti, cioè sulla ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse possibili forme di ammortizzatore sociale, prenda posizione in modo molto chiaro e netto. Su questo attendiamo una risposta del Governo.

quell'emendamento faceva sì che i lavoratori dipendenti o comunque i redditi assimilati al lavoro dipendente potessero avere, in questo periodo di luglio, agosto e settembre, una detassazione sulle retribuzioni.

l'emendamento 4.201 è molto semplice e inquadra la necessità di dare stabilità all'occupazione di molti soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utile presso gli istituti scolastici. C'è un tema vero

di lavori socialmente utili e sono attualmente impegnati negli istituti scolastici, dove svolgono una funzione utile ai fini del mantenimento degli istituti stessi e anche delle normali attività Grazie,

Il rapporto di lavoro tra i medici fiscali e l'INPS è regolato in base alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 463 del 1983, come convertito dalla legge n. Va rilevato che i medici hanno con l'istituto un rapporto fiduciario essendo inseriti in liste speciali. Fermo restando l'attuale tipologia del rapporto libero-professionale e in attesa di una completa rivisitazione della materia mediante la modifica della legge n. 1'ordine del giorno intende confermare la consistenza numerica dei sanitari inseriti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007, come stabilito con il decreto interministeriale dell'8 maggio 2008, si pone come obiettivo di dare un minimo di stabilità lavorativa ai sanitari già incaricati, molti dei quali in servizio presso l'INPS da oltre un decennio, che hanno già ottenuto la conferma dell'incarico nel 2000 e nel 2008, superando l'attuale stato di insicurezza.

con cui si impegnava il Governo «ad adottare le iniziative necessarie per l'adeguamento del quadro normativo che finora ha regolato la specifica materia, così come espressamente indicato nelle premesse del decreto ministeriale dell'8 maggio 2008, per dare certezza ai medici già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007, trasformando le liste speciali, già costituite ai sensi del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 dell'11 novembre 1983, in liste speciali ad esaurimento nelle quali confermare i medici iscritti alla predetta data del 31 dicembre 2007». Chiediamo quindi al Governo Letta di rinnovare tale impegno, preso appena sei mesi fa dal Governo Monti, e di trasformarlo in una disposizione normativa. Un'eventuale rimodulazione della disciplina a legislazione costante, già proposta informalmente dalla stessa INPS, comporterebbe la immediata decadenza dall'incarico degli attuali sanitari, senza alcuna garanzia di un'ulteriore riconferma, la conseguente perdita di professionalità acquisite in tanti anni di servizio. Restando invariata la tipologia dell'incarico e, di conseguenza, l'attuale disciplina che viene regolamentata con decreto interministeriale, l'ordine del giorno in argomento non prevede l'introduzione di alcun onere a carico della finanza pubblica, lasciando ai Ministeri competenti (lavoro e salute) di stabilire, come già avviene, i compensi che sono riconosciuti a prestazione, senza alcun obbligo per l'INPS di assegnazione di un numero determinato di visite da effettuare, attualmente stabiliti dal decreto ministeriale dell'8 maggio 2008. Il provvedimento che proponiamo riguarda i sanitari iscritti nelle liste su tutto il territorio nazionale che hanno un'età media tra i 50 e 55 anni e che, a causa del regime delle incompatibilità, non hanno potuto frequentare le scuole di specializzazione *post lauream* o i corsi specifici in medicina generale e, nel caso di perdita dell'incarico, che per molti rappresenta l'unica fonte di reddito, avrebbero serie difficoltà di reinserimento lavorativo. Quindi, chiediamo al Governo

dell'area ionico-etnea, un'area che traballa: quest'anno abbiamo avuto 52 effetti eruttivi, oltre i rischi eruttivi dell'Etna. Sappiamo che l'Etna, ormai da oltre dieci anni, ha l'abitudine - e lo ha fatto già 35 volte - di dare origine a effusioni sabbiose che provocano danni gravissimi all'economia, alla vivibilità e all'agricoltura della nostra terra. Siamo in una terra, di fronte alla faglia ibleo-maltese,

all'indomani di alcuni fenomeni, cioè di due forti scosse telluriche e di una grande quantità di sabbia che quasi seppellì la provincia etnea, insieme ovviamente ai fenomeni eruttivi,

fino ad oggi, hanno consentito di supportare le amministrazioni locali nei cosiddetti uffici sisma che hanno il compito di monitorare la situazione e i comportamenti del vulcano Etna,

ad ormai oltre dieci anni dall'inizio della loro collaborazione, per l'esperienza maturata in questi Comuni, possano essere stabilizzate, perché è corretto nei confronti di professionisti che hanno dedicato la parte migliore della loro vita a questo tipo di attività, ma perché sarebbe indecente privare i Comuni ad alto rischio dell'area etnea degli uffici sisma e dei professionisti che li hanno sostenuti finora.

Noi dobbiamo considerare questo come un atto prodromico e urgente: prodromico, perché presupposto di quella che poi dovrà essere la ridefinizione del tema complessivo della tassazione immobiliare; urgente, perché è proprio il punto da cui si parte per poter poi proseguire. circostanza che verranno affrontati questi temi anche in sede di indagine conoscitiva ci porta, a fronte dei 42 emendamenti presentati all'articolo 1,

uno *spot* che si inquadra in un più ampio disegno che riguarderà la definizione della tassazione immobiliare. Quindi, invito i presentatori al ritiro di tutti

Anche per gli emendamenti in materia lavoristica prevale l'esigenza di una definitiva conversione in legge del decreto-legge. Pertanto, il parere contrario si associa ad una

a valutare la possibilità di introdurre misure volte a contrastare la povertà estrema, anche portando a regime misure sperimentali già varate con successo negli anni recenti».

a mettere in atto, nei limiti imposti dal rispetto delle sfere di competenza statali e regionali, a mettere in atto

Il senatore Marinello

ringrazio la collega, che ha accolto l'invito che avevo rivolto, a lei come ad altri proponenti,

avvisare il Governo di non produrre disposizioni che sono in contraddizione con le norme di contabilità pubblica. Come si faccia a stabilire che i bilanci preventivi possano essere redatti nella seconda metà dell'anno l'ordine del giorno che impegna il Governo a trattare la vicenda dei bilanci comunali in modo congruo

sul quale, negli anni scorsi, si è un po' lentamente ceduto, sia da parte del Governo sia da parte degli enti locali. La necessità di approvare i bilanci di previsione entro il 31 dicembre dell'anno

sull'osservazione del Patto di stabilità, sui bilanci delle partecipate e su tutta una serie di attività, anche di governo, dell'ente locale, che viene costretto a ricorrere per la maggior parte dell'anno all'esercizio provvisorio, e che quindi non può dimensionare le sue dinamiche anche di governo locale secondo i suoi progetti e secondo le esigenze di finanza pubblica. Quindi credo che su questo dovremmo attivare anche in Commissione bilancio, ma soprattutto, in contraddittorio con il Governo, una normativa per la quale, al classico decreto di proroga del termine per la presentazione del bilancio, si integrino norme per cui i Comuni possono comunque approvare i bilanci in tempo e magari poi, in sede di variazione degli stessi, eventualmente inserire alcune novità relative alle leggi che si vanno proponendo

desidero sottoporre al Governo il problema che spesso, o meglio, sempre, questa pratica, che oramai è diventata quasi consuetudine, di approvare i bilanci preventivi a fine anno, deriva dall'incertezza normativa delle risorse finanziarie messe in campo per cui i Comuni che sostanzialmente devono fare un bilancio rispetto alle norme, ai trasferimenti e al gettito locale non sanno come fare. Però diventa un problema grande, perché poi si lavora per dodicesimi rispetto all'anno precedente e sostanzialmente tutte le amministrazioni comunali sono bloccate.

poter dare ai dirigenti, entro tempi utili, il piano esecutivo di gestione e definire, quindi, tutti gli obiettivi che la struttura deve perseguire. In nessuna azienda privata si danno gli obiettivi nel mese

Il presidente di Confindustria, tre giorni fa, ha detto che se non riparte l'edilizia, non avremo un rilancio del prodotto interno lordo. Siamo tutti d'accordo:

L'emendamento 1.202 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.202.

interesse: come ricorda spesso il senatore Chiti in Commissione politiche comunitarie, bisogna evitare le procedure d'infrazione

Contemporaneamente, ha stabilito la proroga delle concessioni demaniali fino al 2020, in violazione delle disposizioni comunitarie. Quali

a chi già ha ottenuto vantaggi, che il Governo conosce benissimo, sono il minimo che possiamo chiedere proprio per salvare questi soggetti imprenditoriali dalla mannaia della procedura di infrazione dell'Unione europea. Non solo, si tratta anche di regolamentare e coordinare le disposizioni nazionali con quelle che vigono in sede regionale. Allora non capisco per quale ragione, se non per qualche pulsione di tipo corporativo e molto poco nobile,

per cento del nostro PIL e le concessioni demaniali a fini turistico-ricreativi che interessano l'attività di balneazione, ma anche gli ambiti interni, i laghi e i fiumi delle nostre Regioni, hanno rilevanza come valore aggiunto da aggregare ai pacchetti turistici integrati.

e sono d'accordo con il Governo. Infatti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito un tavolo tecnico proprio per adempiere a quell'impegno che il Governo aveva assunto anche nella legislazione precedente a seguito della proroga delle concessioni demaniali al 2020,

(che sono di una gravosità insostenibile per un numero molto importante di imprese turistico‑balneari), un aumento indifferenziato dei canoni del 10 per cento significherebbe

particolare situazione economica che vivono oggi le realtà dell'edilizia e in generale tutte le imprese del tessuto produttivo italiano, soprattutto - lo ripeto - quelle che hanno lavorato in questo settore, credo vada dato un segnale di sensibilità e di attenzione, che non è,

ricordargli che "il Governo in Parlamento" è un'istituzione parlamentare: non riesco quindi a capire di cosa si dolga quando Parlamento e Governo interloquiscono.

apprezzo l'intervento dei colleghi. Non so se siamo nella fisiologia del rapporto tra Parlamento e Governo. Cercavo di ragionare in termini costruttivi su una questione che è fondamentalmente di metodo e che si rifaceva a quello che avevamo detto all'inizio. L'intervento della senatrice Puppato poteva far ritenere che noi la pensassimo diversamente sul merito, ma allora ci siamo spiegati molto male, così come ci siamo spiegati male sulle conclusioni alle quali si stava lavorando in 6a Commissione.

Signor Presidente, ho illustrato prima la bontà degli emendamenti da me presentati ed il loro grande significato rispetto alle tutele che noi dobbiamo saper prevedere per interi settori produttivi, peraltro così significativi, in questo caso, del nostro sistema economico.

anche degli emendamenti 4.9 e 4.200, tutti inerenti al tema che abbiamo provato a sviluppare nella conversione di questo testo e che ci riproponiamo di

sull'oggetto di questi due emendamenti, ritirati o no che essi siano. Stiamo parlando di cassa integrazione, cioè di una forma di provvidenza volta a tenere legati i lavoratori all'azienda da cui dipendono e fondata normalmente su di un rapporto assicurativo. Di regola, la cassa integrazione è attivata per aziende che pagano un contributo all'INPS, nell'ambito di un rapporto di assicurazione. Ora, questi emendamenti mirano a estendere il trattamento di cassa integrazione a un settore - quello degli studi professionali

non si vede per quale motivo si debba estendere a un settore come quello degli studi professionali questa prestazione assicurativa senza che gli studi stessi siano tenuti al versamento del relativo Un conto è far fronte a una situazione di gravissima emergenza con un provvedimento eccezionale e temporaneo; altro conto è, a ben cinque anni di questo strumento eccezionale (quindi in situazione che non può più considerarsi eccezionale e temporanea),

Per altro verso, avverto che il Governo dovrà scegliere tra accogliere la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento Bonfrisco e accogliere come ordine del giorno la trasformazione dell'emendamento 4.20, presentato dal Gruppo di Scelta Civica, perché i due ordini del giorno vanno in direzione diametralmente opposta l'uno rispetto all'altro. In conclusione, chiedo che riflettiamo attentamente su questo problema e che non prendiamo

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vedo invero questa contraddizione, perché già ora la disciplina degli ammortizzatori in deroga (che è, come noto, una disciplina molto flessibile) consente e ha consentito ad alcune Regioni di comprendere anche i dipendenti degli studi professionali. Quando che sono strutture complesse, si trovano di fronte a consistenti cali di fatturato e tuttavia, pensando di poter

non vedo motivo per negare l'utilizzo di uno strumento che è stato concepito nel contesto della grande crisi proprio in funzione di quegli ambiti lavorativi e produttivi che non sono protetti dall'assicurazione obbligatoria. che non sono protetti dall'assicurazione obbligatoria. Questa è la ragione principale degli ammortizzatori sociali in deroga. ad un uso quanto più oculato. Ho parlato per primo, nell'ambito della relazione, di ammortizzatori che sono stati utilizzati

Cosa diversa è l'esigenza di fissare criteri d'impiego di questi strumenti, quale è indicata nell'ordine del giorno

una raccomandazione. Insomma, non vedo ragioni di contraddizione tra la possibilità di accogliere questo ordine del giorno e quella poi di accogliere come raccomandazione quello da lei presentato.

Colgo qui l'occasione per esprimergli riconoscimento per la possibilità che ha dato alle strutture professionali di sfruttare la cassa integrazione in deroga, ovviamente quando queste sono strutture complesse. Si pensi alle strutture sanitarie le quali, per le note vicende dovute ai disavanzi delle Regioni sottoposte ad un piano di rientro dal debito,

un commissario *ad acta*, il dottor Francesco Massicci (che è un po' il cerbero della spesa sociale), taglia le tariffe di remunerazione per le prestazioni sanitarie

viene pagato a pie' di lista. Allora le Regioni cosa fanno? Il Governo crea le condizioni perché si inaspriscano il disagio e la condizione fallimentare delle strutture sanitarie che, ovviamente, accederanno in maggior numero ai proventi e alle possibilità che la cosiddetta legge Sacconi ci consente.

quelli che soggiacciono a questi tagli, e quindi vedono diminuire la qualità e la puntualità dell'offerta sanitaria, sono i malati, i pazienti, sono coloro che ancora oggi si rivolgono alle strutture accreditate che tutti i Governi di questa Repubblica, statalisti e dirigisti quali sono stati, hanno sempre ritenuto una mera appendice a favore di un servizio pubblico che continua ad essere considerato monopolio dello Stato.

il senatore D'Alì aveva già presentato un ordine del giorno che ricomprende, oltre ad altre questioni, la questione specifica del

condivido le sue valutazioni. Mi ritrovo però maggiormente rappresentata da quella scuola di pensiero, professor Ichino, che punta

per nostra consuetudine ed impostazione culturale (prima ancora che politica), abbiamo sempre dedicato al lavoro dipendente (sono senatore Ichino, non sfugga che si tratta di lavoratori dipendenti degli uffici o del settore delle professioni in generale), ad un certo tipo di lavoro dipendente che va riducendosi

Ricordo solo quanto importante sia stato, ad esempio, nel passato, professor Ichino, ampliare a una platea diversa, come quella delle imprese artigiane,

Quindi, nel rispondere alla proposta del Governo, ritiro, certamente, l'emendamento e sottoscrivo l'ordine del giorno G4.2, presentato dal senatore D'Alì, che ricomprende buona parte di questo tema.

Non abbiamo alcuna notizia su come siano ripartiti questi casi tra i settori dell'industria, dell'artigianato e degli studi professionali, ma è più che ragionevole pensare che questo fenomeno sia equamente ripartito fra tutti i settori. Poiché esiste l'assicurazione sociale per l'impiego, cioè un trattamento di disoccupazione che copre per un intero anno la situazione di disoccupazione con contribuzione da parte del datore di lavoro, e poiché questa forma di previdenza si applica anche ai dipendenti degli studi professionali,

Signor Presidente, con l'emendamento 4.6 abbiamo chiesto che, invece di stanziare 250 milioni di euro reperendoli dal Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività, si potessero stanziare 500 milioni di euro a valere sulla previsione di un tetto per le pensioni alte erogate esclusivamente con il sistema retributivo.

Dichiaro aperta la votazione.

un tema che esula dai profili di copertura finanziaria che finora abbiamo affrontato a proposito del settore delle libere professioni e si concentra sulla rappresentanza

la trasformazione in ordine del giorno è anche più congrua rispetto a una rigida norma di legge, in quanto si tratta di relazioni

stiamo parlando di cassa integrazione, quindi di un provvedimento rivolto a sostegno del reddito per lavoratori dipendenti che vengono sospesi dal lavoro per una crisi occupazionale aziendale. Il secondo comma dell'articolo 4 prevede che il Ministro, sentite le parti sociali, emani le istruzioni, le regole, per la ripartizione e l'erogazione della cassa integrazione in deroga. "In deroga", sì, ma sempre di cassa integrazione si tratta, quindi di un provvedimento per sua natura destinato a lavoratori dipendenti.

le parti sociali che possono e devono essere interessate a esprimere un parere sui criteri di erogazione della cassa sono i sindacati dei lavoratori dipendenti.

di vivere: quella del dialogo con le parti sociali in relazione proprio a questa strumentazione straordinaria utilizzata nel tempo di crisi con fini di coesione sociale e di continuità delle attività produttive: attività produttive di beni come di servizi. Il dialogo che le istituzioni intrattengono con le parti sociali - come è noto - riguarda le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro. Tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, firmataria di contratti collettivi c'è un'organizzazione che rappresenta gli studi professionali non in quanto lavoratori autonomi, ma in quanto datori di lavoro; e in quanto datori di lavoro essi sono consultati proprio ai fini dei criteri di erogazione - così è stato in passato e così ragionevolmente sarà in futuro perché la individuazione dei modi più opportuni con i quali impiegare queste risorse passa anche attraverso il confronto con i rappresentanti delle imprese produttrici di beni o di servizi, compresi gli studi professionali, che sono datori di lavoro - prima sono stati citati anche i numeri dei loro dipendenti loro dipendenti - e stanno vivendo una condizione critica anch'essi, come altri ambiti del nostro terziario. Ora, non comprendo queste preoccupazioni perché appartengono, in ogni caso, Grazie onestamente ritenere che le più rappresentative debbano riguardare tutti gli ambiti merceologici - insisto - di beni come di servizi, proprio perché la crisi ha caratteristiche diffuse, generalizzate. Quindi, pur rispettando tutte le

fosse accolta dal Governo come ordine del giorno. Si tratta di fare esattamente quello che saremo costretti a compiere. Siccome le dotazioni finanziarie della cassa integrazione in deroga sono inadeguate,

Dichiaro aperta la votazione.

l'ordine del giorno G4.20 può essere accolto come raccomandazione poiché indica i criteri di concessione che, peraltro, saranno oggetto di un decreto ministeriale, sentite le parti sociali, le Regioni e le Commissioni parlamentari. Quindi, avremo modo di discutere dei criteri stessi prima che vengano approvati attraverso uno strumento di normazione secondaria.

gli obiettivi che si propongono sono condivisibili perché riguardano una gestione più attenta e più coerente con la lettera la lettera e lo spirito della legge che vorrebbe gli ammortizzatori sociali dedicati quanto più alla continuità del rapporto di lavoro e ad un doveroso accompagnamento anche con cosiddette politiche attive, che spesso sono state carenti.

al risultato che chiede il relatore, perché esso è formulato nel senso di impegnare il Governo a tener conto dei criteri indicati nell'emendamento: questo implica

di questo fenomeno, ma anche il contenimento dell'espansione su questo settore di fenomeni di criminalità organizzata, noi ritireremmo l'emendamento.

Dichiaro aperta la votazione.

procedure di stabilizzazione del personale assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali atipiche in modo tale che non ci sia una articolazione per settore o per ambito territoriale regionale un po' troppo varia, per cui alcune alcune procedure di stabilizzazione sono portate avanti, altre vengono dimenticate, in alcune si riconosce il servizio prestato, in altre non lo si riconosce. Si tratta di operare, ove

Dichiaro aperta la votazione.

Proprio perché consideriamo il merito, e non c'è differenza di approccio da parte del relatore (e credo ugualmente da parte del Governo), purtroppo l'ordine del giorno G4.3 a una specifica limitazione delle risorse, che dovrebbero affluire agli ammortizzatori sociali in deroga, che non può essere accolta,

risaltano gli ex lavoratori delle Case di cura riunite di Bari i quali, dopo 18 anni - ripeto: 18 anni - di ricorso agli ammortizzatori sociali tra cui la cassa integrazione in deroga, non hanno ancora avuto una diversa ricollocazione lavorativa;

a promuovere presso la Regione Puglia l'individuazione di enti strumentali cui affidare attività riferibili alle competenze maturate» da questi lavoratori nelle Case di cura in 18 anni di non-lavoro. Mi chiedo quale paziente possa affidarsi alle competenze professionali maturate in 18 anni di cassa integrazione, in deroga o non in deroga che sia. Questi dati sono la certificazione del fallimento di un intero sistema di ammortizzatori sociali, di un intero sistema con cui si affrontano le crisi occupazionali nel nostro Paese. Se continuiamo a trastullarci con le proroghe di questi strumenti condanniamo il Paese a rimanere in una situazione di cronica inferiorità! Diciamo allora le cose come stanno: 18 anni di cassa integrazione sono 18 anni di una menzogna, cioè di finzione dell'esistenza di un posto di lavoro che non c'è. Sono quindi 18 anni di abuso di uno strumento che non potrebbe essere utilizzato nel caso abuso che fa sì che il lavoratore resti in questa posizione per 18 anni invece che essere aiutato a trovare una nuova occupazione. Non nella casa di cura ex-datrice di lavoro, che evidentemente non esiste più: non è quella che può ridargli il lavoro, ma in altri settori. Per questo, occorrono procedure di riqualificazione professionale e incentivi perché il lavoratore si attivi; noi invece mettiamo in atto incentivi perché il lavoratore non si attivi e resti per 18 anni in attesa passiva. Allora chiedo al Governo:

il caso delle Case di cura riunite di Bari è invero una vicenda, per fortuna, pressoché unica nel Paese. Ed è pressoché unica, perché ha caratteristiche che andrebbero davvero indagate, sotto vari punti di vista, per come quella vicenda è nata, si è sviluppata e si è trascinata nel tempo. Meriterebbe davvero attenzione, ed ho visto applausi provenienti anche da banchi che dovrebbero far riflettere sul percorso e sulle responsabilità di questa vicenda. In ogni modo, quanto dice il senatore Ichino è assolutamente giusto: è una situazione che non può dare luogo a una infinita proroga degli strumenti tradizionali

come sempre - quando si depositano responsabilità colpevoli delle amministrazioni pubbliche, che hanno così generosamente nel tempo accompagnato questa vicenda, e si sono determinate nelle persone condizioni di attesa di una soluzione che nel frattempo non è stata organizzata nei termini corretti, è ovvio ovvio che la funzione pubblica debba guardare a quel caso ed individuare modalità specifiche, proprio per ciò che si è depositato nel tempo rispetto a terzi incolpevoli, che non possono essere associati alle responsabilità pubbliche. Questa è la caratteristica di questa vicenda, che mi ha visto più volte personalmente molto critico verso di essa. In questo senso, l'accoglimento come raccomandazione di questo ordine del giorno avrebbe potuto sollecitare il Governo ad un'attenzione con modalità diverse da quelle tradizionali. Ma, ciò detto, per quanto mi riguarda, il massimo di accoglimento poteva essere una raccomandazione nel senso che ho espresso; altrimenti,

del giorno mette una toppa ad un buco ancora più grande che l'intervento del relatore aveva creato, perché, come sempre accade, veniamo chiamati a svolgere un ruolo da chi quel ruolo forse ha avuto l'autorità e anche l'incarico per poterlo risolvere negli anni passati. Comunque, visto che c'è il ritiro dell'ordine del giorno, stendiamo un velo pietoso su una vicenda che che peraltro impegnava il Governo non ad assumere iniziative proprie, ma a rimandare alla Regione Puglia la ricerca di enti strumentali cui affidare questi lavoratori. Credo che il ritiro metta una toppa ad un'altra vicenda singolare. PRESIDENTE. Era un tentativo di sussidiarietà, evidentemente.

a tutela sia delle amministrazioni che dei lavoratori. Tuttavia, per anni sono stati costretti ad accettare in modo coatto l'esclusività professionale, e quindi - oggi si trovano nell'impossibilità di accedere ad altre esperienze professionali. Quindi, invitiamo il Governo a trovare soluzione a questo problema, che altrimenti rischia di diventare unico come

l'articolo, l'ennesimo pasticcio burocratico fiscale, che mette a rischio la sopravvivenza stessa di gran parte dell'economia etnea, può essere risolto solo dalla politica. A fare questa affermazione, e ad anticipare un emendamento sul "decreto del fare" che verrà al Senato,

ministri del 2002 prevedeva, da una parte, attenzioni a quelli che erano i problemi economici derivati dai danni delle ceneri vulcaniche e dal sisma, oltre che dai danni eruttivi dall'altra, una organizzazione di tutela dei Comuni che monitorasse e prevenisse questa condizione. Adesso noi abbiamo un Ministro di formazioni politiche diverse, ma ovviamente impegnati insieme nel Governo, che si impegnano a fare retrocedere il fisco, che sta chiedendo il 50 per cento dei contributi compensativi all'economia della Sicilia in quell'ambito, e dimentichiamo, invece, di valutare, signora Sottosegretario, la necessità che gli uffici sisma che operano da 11 anni nei Comuni e che impegnano, come ho ribadito, 29 supertecnici tra ingegneri, architetti e geologi, possano continuare a tutelare un territorio ogni giorno gravemente a rischio,

è d'uso, sono sempre in coppia, o perché rappresentano le due parti politiche tra loro contrastanti e contrapposte o perché sono chiamati ad affrontare i temi dei decreti-legge predisposti dal Governo in più Commissioni, proprio perché il loro contenuto è disomogeneo, non organico organico rispetto alla funzione principale cui dovrebbero assolvere i decreti-legge. I decreti-legge dovrebbero avere carattere d'urgenza, dovrebbero trattare questioni assolutamente indifferibili e dovrebbero mettere il Paese nelle condizioni di affrontare delle emergenze che, come sembra ovvio considerare, devono avere un carattere di straordinarietà. Se noi rimaniamo in una condizione di emergenza

se a farlo cadere sarà una disattenzione di qualche Ministro, oppure problemi più consistenti di politica estera. estera. Sta di fatto che siamo di fronte ad una condizione che richiamerebbe l'esigenza di andare a votare subito per tentare di fare chiarezza.

Governo, e che sono chiamati ad esercitare la loro funzione per quanto riguarda l'imposta sugli immobili, in modo particolare una sospensione dell'imposta sugli immobili per alcune categorie di soggetti e alcune categorie di abitazioni. Questa partita, ci dice il ministro Saccomanni, verrà ripresa integralmente entro il mese di agosto, e su questa partita la Commissione finanze ha attivato una procedura conoscitiva per capire come deve essere articolata la fiscalità sugli immobili,

per i lavoratori espulsi dal sistema produttivo. Ricordo al senatore Ichino che non parliamo di 10, 20, 100, 500.000 lavoratori facilmente reinseribili all'interno di un sistema economico sano: sono, purtroppo - ci ha annunciato il ministro Giovannini - 6 milioni, e stanno dentro un sistema economico malato, incapace di reagire. La terza questione che viene trattata in questo provvedimento è una sorta di proroga del lavoro precario, sviluppatosi precario, sviluppatosi a causa di un blocco delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, blocco che viene puntualmente derogato perché comunque devono essere resi alcuni servizi.

modo l'obiettivo di rendere meno sofferente la condizione di alcune categorie particolarmente in difficoltà, cioè i cittadini possessori di prima casa, molti dei quali sono in trattamento previdenziale - e quindi pensionanti - e molti altri sono lavoratori dipendenti o piccoli imprenditori, quindi persone che vivono con redditi misurati; altri sei mesi di attività lavorativa per coloro che vivono una condizione di precarietà. Per tale ragione, cioè per il piccolo passo che si compie verso la sofferenza,

di una modalità di gestione del declino del nostro Paese, su cui le forze politiche con maggiori responsabilità e maggiori consensi si stanno

su suggerimento di un Governo che dovrebbe essere favorevole al libero mercato e che invece contraddice se stesso, la sua funzione, la sua provenienza politica semplicemente per fare una sorta di piacere ad di piacere ad una *lobby* corporativa che ha interesse a mantenere chiuso quel mercato.

Grazie

il Governo ha dato le indicazioni nella giusta direzione e pertanto trova condivisione.

noi non abbiamo votato la fiducia al Governo per gestire un declino, per avere una dolce morte della nostra economia e un dolce appiattimento verso i centri di potere dell'economia mondiale o europea; di certo abbiamo dato fiducia all'attuale Governo, e oggi siamo contenti di averlo fatto, perché crediamo che questo Governo e questa larga maggioranza che lo sostiene rappresentino la ricetta migliore per combattere il lento declino, determinato anche da posizioni sempre di contrapposizione troppo nette, troppo decise e troppo influenzate dalla propaganda. Anche nell'ultimo intervento, il senatore Uras quasi ci chiamava alla soddisfazione che ne potrebbe trarre politicamente da da un indietreggiare della nostra economia o della nostra occupazione. No, noi siamo per la cultura del fare; noi siamo per la cultura della prospettiva, della speranza, perché oggi è criminale chi toglie la speranza alle nuove generazioni. Oggi chi non si accorge, chi è troppo sordo e cieco per capire la disperazione delle nuove generazioni davvero si assume una grande responsabilità. Non possiamo dividerci; non possiamo issare stendardi ideologici

chi non è cattolico sa che la laicità, il comportamento, il fare sono doveri di chiunque voglia assumere la rappresentanza. Oggi è il tempo del fare, oggi è il tempo di dare risposte. Certo, non contingenti, come quelle che stiamo proponendo oggi: oggi, lo sappiamo, cerchiamo di tamponare una crisi per avere riforme strutturali a settembre, a ottobre, il più presto possibile. Oggi sapevamo che dovevamo bloccare il pagamento dell'IMU, perché era un'offesa, e ve lo dico da uomo del Meridione. Chi si costruisce la casa nel Meridione non lo fa per avere uno *status symbol*, per dimostrare di aver raggiunto la ricchezza o il successo sociale ed economico; chi costruisce la casa nel Meridione lo fa dando risposta a un sentimento antico, indatabile, che si alla capanna, alla grotta, al rifugio. L'ambizione più grande di un genitore del Mezzogiorno d'Italia è quella di poter fare lo stesso per il proprio figlio. intesa come bene riparo, come il tutto di una vita lavorativa e anche di sentimenti, non poteva essere l'oggetto principale della tassazione, non poteva continuare a essere l'oggetto cupido cupido delle nostre entrate, pertanto la si blocca, e si determina un nuovo corso, un ridisegno. Appoggiamo pienamente, siamo d'accordo e sosteniamo il Governo quando ci dice che affronterà in maniera organica il ridisegno di questa imposta, quando si rivedranno queste tematiche. Ringrazio il sottosegretario De Camillis che, a nome del Governo, ha accolto il nostro ordine del giorno G1.100 (testo 2) su un altro aspetto di questa odiosa tassa, che, quando va a colpire settori già in crisi, determina un'ulteriore ingiustizia. Infatti, è bene che si tassino le attività che producono reddito; è bene che paghino le tasse tutti coloro che hanno benefici o rendite; è bene che ci sia la giustizia fiscale e quindi sociale, e che la si raggiunga in tutti i settori; tuttavia, quando questo non è più possibile, quando sembra quasi che l'atteggiamento del fisco sia quello di tirar sangue da chi ormai è esangue, anemico e non riesce più a dare nulla, allora è lì che va corretto il tiro. Ringraziamo il Governo per averlo fatto oggi nei confronti del nostro Gruppo e degli e degli amici degli altri Gruppi che hanno voluto sottoscrivere il nostro ordine del giorno volto a considerare bene magazzino gli invenduti delle nostre imprese di costruzione. In questo sforzo In questo sforzo per costruire un'Italia dove sia bene poter vivere, dove si possa immaginare il proprio futuro, noi ci saremo sempre. Signor Presidente e cari colleghi,

fatto questo, cari amici, avremo bisogno tutti di vedere le grandi strategie del nostro Paese. Questo andare a ramengo ricercando quali possono essere punti di forza dell'economia non possiamo più consentirlo. mi auguro che al più presto questo ramo del Parlamento possa essere investito delle strategie di crescita, che non possono non vederci protagonisti della più ampia politica europea. Ed è per questo che, anche in senso di sostegno a ciò che il presidente Letta sta realizzando in Europa, daremo convintamente il nostro voto a favore. Signor Presidente, rappresentanti del Governo - ai quali chiedo cortesemente attenzione - onorevoli colleghi, siamo dunque giunti alle dichiarazioni conclusive su questo provvedimento noto a tutti come decreto sulla sospensione dell'IMU. Nonostante, infatti, il provvedimento contenga al suo interno importanti disposizioni anche in materia di lavoro, noi tutti lo conosciamo come il decreto-legge sul rinvio di quella che sarebbe dovuta essere una imposta municipale. municipale. Nel titolo, o per meglio dire, nel suo appellativo, si fa rientrare uno dei provvedimenti più invisi dagli italiani, l'IMU, votato a grandissima maggioranza dal precedente Governo, e il più classico metodo italiano per tentare di risolvere il problema, ovvero il rinvio. E del resto, se il metodo di tartassare i cittadini con nuove gabelle, facendole raccogliere dai sindaci, così da evitare facili e preventivabili critiche, e il continuo posticipo della risoluzione del problema, hanno sempre funzionato, quindi perché cambiarli Per parafrasare il nome di un altro recente provvedimento governativo, potremo allora chiamarlo "decreto del rinviare". Ora però che i conti non tornano più, che i nodi arrivano tutti al pettine, il Governo ci presenta questo provvedimento. proprio dall'analisi della sospensione del versamento della rata di acconto sull'imposta municipale propria, la cui scadenza era fissata lo scorso 16 giugno e che si applicava alle prime case, ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali. Già qui il Governo dimostra tutta la sua mancanza di coraggio, escludendo dalla sospensione anche i fabbricati classificati come categoria catastale D, cioè i fabbricati strumentali delle imprese. Imprese che, come tutti purtroppo sappiamo, sono sempre più in difficoltà, imprese che quotidianamente chiudono. Su questo punto ritengo doveroso, onorevoli colleghi, soffermarmi. Per tanti ragioni. Anzitutto riteniamo incoerente andare ai convegni delle associazioni di categoria, incontrare gli industriali, gli artigiani, promettere a tutti di sostenere la ripresa economica e poi, alla prima occasione utile, cioè questa occasione, dimenticarsi delle aziende e di una delle imposte più inique che su loro grava. E nemmeno un provvedimento per bloccare, o perlomeno sospendere, l'aumento del moltiplicatore relativo agli immobili e ai fabbricati in categoria D, che passa, sempre in virtù di quel celebre decreto salva Italia (che purtroppo l'Italia non ha salvato), da 60 a 65. Un'imposta, tra l'altro, che non è nemmeno municipale. Perché, forse qui qualcuno non lo sa o si è dimenticato, da quest'anno quest'imposta porterà l'intero gettito degli immobili di categoria catastale D allo Stato centrale,

O possiamo ancora sostenere che l'autonomia finanziaria degli enti locali sia uno degli obiettivi di questo Governo? Non parliamo, poi, del rilancio dell'economia o del sistema produttivo italiano.

notare come il provvedimento superi tutte queste incertezze, prospettando una complessiva riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare, nella quale, oltre all'IMU, dovrà essere rivista anche la tariffa sui rifiuti. Ma tutta questa riforma dovrà avvenire - ricordiamocelo - nel «rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 ed in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo». È quindi un margine di operatività, per questo Governo e per il Paese, praticamente nullo, ulteriormente peggiorato dalle nefaste negative previsioni di crescita del DEF stesso piuttosto che dal Fondo monetario internazionale. In realtà, vi sono spazi di manovra per raccogliere quelle risorse necessarie per rivedere l'imposizione immobiliare, e sono anche noti ai membri di questo Governo. Sì, perché l'elusione fiscale, anche e soprattutto in campo immobiliare, sottrae importanti risorse che, viceversa, potrebbero essere destinate a finanziare una tassazione più leggera.

Il provvedimento, così come formulato, risulta caratterizzato da una logica emergenziale e privo di una visione strategica e programmatica, incapace di fornire ai cittadini prospettive di medio e lungo periodo nel segno di una complessiva incertezza sugli interventi e le coperture. Le premesse coraggiose formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri nel suo discorso di insediamento - lo abbiamo tutti ascoltato - si sono rivelate puro fumo negli occhi, considerate le misure contenute nel presente decreto-legge. Sono interventi palliativi, onorevoli colleghi, che tamponano situazioni di impellenza rinviando semplicemente il problema, nessuna azione strutturale volta ad alleggerire il carico fiscale su cittadini, imprese e lavoratori Ma il tempo stringe e la ripresa economica stenta a ripartire. Da tre anni il saldo tra natalità e mortalità delle aziende italiane continua ad essere negativo. Gli ultimi dati ci confermano che, nel primo trimestre di questo anno, la crisi ha fatto chiudere - fate memoria di questo numero - 31.351 imprese, il peggiore saldo dal 2004, e credo che questo debba farci riflettere e non poco.

dall'altro lato è evidente che il Paese e le sue aziende non possono continuare a sostenere una tassazione e un quadro normativo pesante, troppo pesante. Su questo punto noi, Lega Nord, continueremo sempre a lavorare esortando il Governo ad adottare iniziative concrete per rilanciare il Paese, monitorando l'azione concreta, finora debole o inesistente, di questo Governo. Presidente, i senatori dal Gruppo Scelta Civica voteranno a favore di questo provvedimento, ma lo faranno carichi di dubbi e perplessità. Ci lascia infatti perplessi, in primo luogo, la sospensione temporanea del pagamento dell'IMU, decisa in pratica alla cieca, sia per quanto riguarda la copertura finanziaria, perché si fa un'operazione di mera cassa, sia per quanto riguarda la nuova disciplina dell'imposta, di cui non si comincia neppure ad intravedere l'approdo definitivo. Tutto questo più per rispondere alle ragioni di propaganda politica di uno dei partiti della maggioranza che non ad una valutazione circa le priorità che in questo momento possono aiutare a contrastare la dura crisi che stiamo attraversando. Se è infatti vero che la sospensione dell'IMU alleggerisce il carico fiscale sulle famiglie in un momento in cui si registra un forte calo dei consumi, è altrettanto vero che lo stesso risultato si sarebbe ottenuto - e a nostro avviso si dovrà ottenere operando sul cuneo fiscale e tagliando le tasse sull'impresa, a cominciare dall'IRAP che grava sul monte salari. In un quadro di finanza pubblica complesso quale attuale ogni riduzione fiscale deve essere operata in modo da massimizzare gli effetti sulla crescita, stimolare gli investimenti, incentivare le nuove assunzioni. Da questo punto di vista l'IMU serve a poco. Ma c'è di più: se è vero che la proprietà della casa è in Italia molto diffusa, è altrettanto vero che le gravi anomalie della classificazione degli immobili e della determinazione dei valori catastali producono una distribuzione dell'imposta molto spesso difforme dal reale valore degli immobili, realizzando così notevoli iniquità tra i contribuenti. Per di più, solo in pochi casi l'agevolazione fiscale sulla casa riguarda i giovani, che, come noto raramente possiedono una loro abitazione: quei giovani che, a parole, tutti dichiarano di voler aiutare e che regolarmente vengono penalizzati dalle misure adottate. un intervento dell'IMU, che a regime si ipotizza ancor più ampio di quanto non si preveda in questo decreto, avrà anche l'effetto di mettere definitivamente in crisi l'impianto del federalismo fiscale, che molti di noi hanno aspramente criticato, man mano che veniva prendendo forma nella scorsa legislatura nelle mani dei ministri Calderoli e Tremonti, e che oggi dimostra il definitivo fallimento della magica formula tremontiana: vedo, voto, pago. Il federalismo e il suo finanziamento attraverso un potenziamento dei poteri locali di imposizione fiscale hanno generato - come dimostrano i dati pubblicati ieri da «Il Sole 24 Ore» - un'esplosione delle entrate fiscali regionali e locali aumentate dal 1992 ad oggi di oltre il 500 per cento, a fronte di un aumento delle entrate statali, nello stesso periodo, di circa il 95 Un federalismo che producendo duplicazioni di funzioni e moltiplicazioni di apparati burocratici ha tradito tutte le promesse di semplificazione, di riduzione dei costi, di responsabilità e *accountability*, determinando al contrario un aumento del peso della burocrazia e della politica e un incremento vertiginoso della tassazione regionale e locale: tanto che nell'ultimo decennio risulta quasi triplicato il peso delle addizionali locali gravanti sui salari. Quando si affronterà il tema dell'IMU che in Italia, come in tutti i Paesi sviluppati, dovrebbe essere il pilastro della finanza locale, bisognerà avviare anche una riflessione sul federalismo e sull'urgenza di rivedere profondamente un'organizzazione del sistema multilivello divenuta insostenibile sul piano dei costi finanziari, economici e sociali. le nostre perplessità riguardano anche la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga: anche se nell'immediato un loro finanziamento è stato necessario per non far venire meno in un momento di crisi misure di sostegno al reddito, è però altrettanto necessario, ed anzi indispensabile, almeno iniziare a introdurre forme diverse di accompagnamento dei lavoratori nei processi di ristrutturazione del nostro apparato produttivo. Il collega Ichino ha più volte sottolineato come i dati dimostrino che l'istituto della cassa integrazione è ormai sostanzialmente snaturato, perché solo in casi rarissimi il lavoratore rientra nell'azienda da cui è stato sospeso, e i dati evidenziano che quanto più è lungo il periodo di cassa integrazione tanto più si allontana la possibilità di ripresa del lavoro. di ieri il dato fornito dal presidente dell'INPS secondo cui negli ultimi quattro anni lo Stato, tramite l'INPS, ha erogato circa 80 miliardi di euro di cassa integrazione e di indennità di disoccupazione a circa tre milioni di lavoratori all'anno: un fiume di denaro che non ha aiutato i lavoratori a formarsi per essere pronti a un mercato del lavoro che chiede nuove professionalità, un fiume di denaro che ha sottratto opportunità di lavoro, possibilità di far crescere l'attività delle aziende e che non ha reso dinamico un mercato del lavoro la cui rigidità è una delle principali ragioni di scarsa attrattività degli investimenti industriali in Italia. Insomma, in un'epoca di trasformazioni profonde dei settori e dei modi di produrre, gli ammortizzatori attuali finiscono per essere una trappola mortale da cui è difficile uscire per rimettersi nel mercato del lavoro e il rinvio a settembre della trattativa con le parti sociali deciso ieri dal ministro Giovannini non è certo un segnale incoraggiante da questo punto di vista. Questo decreto si muove comprensibilmente nella logica dell'emergenza: l'emergenza del lavoro e quella - lasciateci dire - dell'irragionevolezza della politica. Ci saremmo però aspettati che contenesse un sia pur timido segnale nella direzione del cambiamento. L'assenza di un tale segnale ci preoccupa, perché solo una diminuzione stabile e strutturale del costo del lavoro, da una parte, e un efficiente mercato del lavoro, dall'altra, rimetteranno in moto gli investimenti, la crescita, il lavoro. Il Governo deve guardare oltre l'emergenza o l'Italia non ce la farà. Noi di Scelta Civica siamo in questa maggioranza per fare le riforme e per farle presto, perché non vorremmo che la ripresa arrivasse e il nostro Paese non fosse pronto a coglierla. Se ciò accadesse, sarebbe difficile poi colmare la distanza che ci separa dai Paesi del Centro e Nord Europa. Ma tutto questo sta nelle nostre mani, nella nostra capacità di trasformare la stagione delle larghe e strane intese nella stagione delle riforme. Per ora in questo decreto non ve ne è traccia. Il nostro voto favorevole è quindi un atto di fiducia che ci auguriamo il Governo apprezzerà e che, soprattutto, non vorrà tradire e deludere.

ancora una volta ci ritroviamo a dover esprimere il nostro voto su un provvedimento minestrone, in cui sotto il ricatto dell'emergenza si mescolano materie tra loro differenti. Non è atto politico, perché risulta totalmente privo di ogni visione strategica ed incapace di fornire prospettive di medio e lungo periodo. Se è un ponte, è un ponte verso il nulla: nessuna azione strutturale volta ad alleggerire il carico fiscale, nonostante il tempo stringa e la ripresa economica fatichi a ripartire. Si persevera nell'unica attività attività politica in cui questo Governo e questa maggioranza sembrano eccellere: rinviare e prevedere solo azioni tampone con incertezza sugli interventi e sulle coperture. Eppure, non sono passati anni da quando il presidente Letta venne a chiedere la fiducia promettendo scelte coraggiose e la centralità del Parlamento, ma al posto di quei proclami continua nel gioco degli specchi e i Sottosegretari vengono in Commissione a chiedere la blindatura dei provvedimenti con la scusa dell'emergenza. È un ritornello che sentiamo ripetere da oltre vent'anni. Attraverso essa anche questo Governo, coerentemente con quell'intreccio di potere che sinora ha gestito la cosa pubblica come se fosse cosa propria, continua a chiedere agli italiani di tenere la schiena curva e di sopravvivere in una bolla di precarietà artificiale, in cui l'abuso degli ammortizzatori sociali è *elisir* di lunga vita di una classe politica e sindacale divenuta parassitaria; è una sovvenzione occulta alle imprese-scatole cinesi, una sottrazione di pubbliche risorse senza nulla costruire, secondo lo schema per cui i profitti sono privati mentre le perdite vengono poste a carico della collettività. Ai *mass media* poi è riservato il lavoro sporco: diffondere in modo utile e controllato il panico, per un sistema di scambio ormai ben collaudato nel mantenere in vita questo *status quo*. La politica degli ultimi decenni, invece di parlare di uguaglianza, di solidarietà, di innovazione, ha inventato la parola magica: emergenza. Siamo in una situazione in cui la classe media sta lentamente ma inesorabilmente scivolando verso la soglia della povertà ed in cui cento della popolazione detiene oltre il 45 per cento della ricchezza, oltre tre milioni di italiani vivono nella povertà assoluta, il 17 per cento degli italiani ha un reddito al di sotto della soglia di povertà e un giovane su tre è senza lavoro e gli altri due sono precari o soggetti a *dumping* salariale. Le politiche di sviluppo nazionali avrebbero dovuto favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione e invece hanno causato soltanto delocalizzazione e drammatica disoccupazione. E invece gli atti politici? Oggi rinviamo l'IMU, domani forse l'IVA, ieri la TARES, senza avere il coraggio di trovare soluzioni definitive alla crisi economica che attanaglia, che è anche nel mondo del lavoro e che richiederebbe una revisione delle politiche passive in favore delle politiche attive, in grado di diminuire il peso del fisco e di alimentare l'occupazione per ridare dignità ai cittadini. Ma c'è l'emergenza, ci dicono, bisogna tenere i conti a posto perché è l'Europa che ce lo chiede. Se così fosse - e ne dubitiamo - sarebbe arrivato il momento di concludere che gli interessi di alcuni Paesi dell'Unione europea cominciano a non essere coincidenti con i nostri. L'Italia, Paese fondatore di questa Europa unita, deve chiedere di poter uscire da quest'*impasse* con dignità uguale agli altri popoli europei. La moneta unica - immaginario strumento per accelerare l'unione politica - è stata pensata è perseguita nell'illusione che non ci sarebbero mai state crisi finanziarie e men che mai crisi politiche, non risultando nemmeno prevista la possibilità di uscita dall'euro. Invece la crisi è arrivata ed è diventata crisi dei debiti sovrani e, dopo la cura da cavallo, siamo ormai ad oltre 40 imprese che falliscono ogni giorno, con un debito pubblico

sono dati della Banca d'Italia - nel primo trimestre sono ulteriormente aumentate dell'1,7 per cento, con una riduzione del PIL del 2,4 per centro rispetto allo stesso periodo del 2012 e dello 0,6 per cento rispetto al semestre precedente, attestandosi la pressione fiscale, stima del Tesoro, oltre il 44,5 Invece di essercene allontanati, siamo paurosamente più vicini all'orlo del precipizio e, se è pur vero che l'uscita dall'euro rappresenterebbe un salto nel buio dagli esiti imprevedibili per un Paese come il nostro che non ha materie prime, stare nell'euro in queste condizioni, senza più un sistema produttivo, comincia ad essere un suicidio. Come abbiamo chiesto nel nostro Documento di economia e finanza alternativo - in cui si è esposta la nostra proposta di governo dell'economia - o si creano strumenti che consentano di dividere il rischio Paese su tutta l'area euro, con la BCE che diventa prenditrice di ultima istanza, o si ristruttura il debito pubblico, congelando il capitale e rinegoziando il tempo di pagamento degli interessi. Questo è già accaduto per la Germania al momento della sua riunificazione, si sta verificando per la Francia e dovrà avvenire anche in Italia, naturalmente con la contemporanea e non più rinviabile revisione delle

Noi parlamentari del Movimento 5 Stelle, solo pochi giorni fa, riducendoci l'indennità alla cifra lorda di 5.000 euro e restituendo quanto non rendicontato della voce diaria, abbiamo restituito allo Stato ben 1,5 milioni di euro. È un'operazione che, se messa in atto da tutti i parlamentari, comporterebbe un ulteriore risparmio di 500 milioni di euro. Per non parlare del fatto che nessun intervento si è avuto il coraggio di fare per imporre il divieto del cumulo anche a quei dirigenti dello Stato che arrivano a percepire retribuzioni Che dire, poi, delle pensioni d'oro? Occorre coraggio e altruismo. Il nostro è un grido d'amore per l'Italia e l'Europa dei popoli. O l'Europa acquisisce consapevolezza che non è più solo e soltanto un mercato ma unione di uomini liberi, e ci si attrezza con una comune rete di salvataggio, equa e solidale, senza ulteriori nodi scorsoi come i vari «*six pack*» e «*two pack*», o la crisi eroderà dalle fondamenta quell'Europa di pace che i vari Adenauer, Churchill, De Gasperi, Schuman e Spinelli avevano immaginato, ridiventando una terra La storia dell'Europa, colleghi, anche quella recente dei nostri nonni, è stata dolorosa e piena di contrasti e sbandate estreme. È però anche storia di un continente che ha visto la culla del progresso e del riscatto degli uomini dalla miseria e che li ha portati al governo del loro destino attraverso la nascita delle costituzioni e del suffragio universale, ora sotto attacco di istituzioni finanziarie come la J. P. Morgan. Quel mondo che fino ad oggi abbiamo conosciuto è in pericolo mortale per le ingiustizie e gli abusi, sociali economici economici ed ecologici. Abbiamo bisogno di una visione costruttiva che sia capace di edificare un nuovo futuro, che è un futuro di senso di comunità, di destino comune. Per fare questo abbiamo bisogno di ambizione, di coraggio e di fiducia in noi stessi. Non bisogna cadere nell'illusione di chi pensa che le cose si aggiusteranno da sole, né nel pessimismo di chi crede che non ci sia nulla da fare. Dobbiamo essere coraggiosi ed ambiziosi e, come diceva Hessel, non dobbiamo arrenderci. Noi del Movimento 5 Stelle siamo qui per rivendicare il diritto del popolo italiano ad avere speranza ed anche se il tragitto è difficile ed impervio, pur nella perdurante diffidenza più totale verso le politiche e le non-scelte messe in atto da questo Governo, voteremo comunque responsabilmente sì a questo disegno di legge, ma continuiamo ad invitarvi ad utilizzare i suggerimenti contenuti nel nostro DEF. I lampi ed i tuoni di tempesta si sentono ancor fragorosi in lontananza e la traversata verso l'approdo sicuro è ancora lunga e se questi nocchieri non sono capaci di affrontarla, perché con lo sguardo chino continuano a rappezzare falle allo scafo da loro stesso procurate o a genuflettersi davanti a capitani stranieri non coraggiosi, è meglio che velocemente lascino il timone a chi non ha paura dei marosi e non chinino la testa:

*(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario De Camillis, arriva alla votazione dell'Aula un provvedimento che è stato tra i primi all'attenzione del nuovo Esecutivo e che è di interesse particolare per il Popolo della Libertà. Esso si inserisce nel quadro delle diverse misure di carattere straordinario emanate nella forma della decretazione d'urgenza per fronteggiare il periodo di straordinaria crisi economica che ha colpito il tessuto produttivo del Paese ed ha impoverito le famiglie italiane. Rientrano in quest'ambito anche il decreto sul pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni alle imprese, il cosiddetto decreto del fare, e le misure per la promozione dell'occupazione (cosiddetto pacchetto lavoro giovani), questi ultimi ancora all'esame delle Commissioni parlamentari dei due rami del Parlamento. Presso le Commissioni finanze e lavoro, che hanno esaminato il provvedimento al nostro esame, si è da subito registrata un'unanime volontà di procedere speditamente all'approvazione del decreto-legge, in pieno accordo con le dichiarazioni dei sottosegretari Baretta e Dell'Aringa; ciò in considerazione dell'eccezionalità della situazione finanziaria della necessità, in particolare, di liberare le risorse, nei rispetto dei vincoli di bilancio imposti in sede di Unione europea, affinché le Regioni potessero utilizzarle per gli ammortizzatori sociali in deroga. In pratica, l'impianto normativo di questo decreto, composto di cinque articoli, consta di tre ambiti: quello tributario, che dispone la sospensione del pagamento dell'IMU sulla prima casa; quello relativo ai contenimento delle spese della politica, e l'ambito più direttamente afferente ai temi del lavoro, che ricomprende il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, i contratti di solidarietà e quelli di lavoro a tempo determinato. Quanto all'ambito tributario, si prevede agli articoli 1 e 2 il rinvio dei pagamento della prima rata dell'IMU, permettendo ai Comuni, considerato il mancato gettito, di ricorrere ad un'anticipazione di tesoreria. La particolare valenza della disposizione va inquadrata nell'ottica di una riforma organica della fiscalità immobiliare, che il Governo intende presentare entro il 31 agosto. Si tratta di una riforma fortemente attesa tutte le famiglie italiane che, spesso con grandi sacrifici, sopportano gli oneri dell'abitazione principale; è perciò fortemente sentita dal Popolo della libertà, che ha sempre sostenuto la profonda ingiustizia sociale e la sostanziale iniquità di una tassazione riguardante la prima casa, facendo del superamento di essa una delle proprie principali battaglie sul piano politico e parlamentare. Altra disposizione che il nostro Gruppo ha giudicato con favore è rappresentata dall'articolo 3, che sancisce il divieto di cumulo del trattamento economico sia per i parlamentari che assumono incarichi di Governo che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si trovino nella medesima condizione. In un periodo in cui il tema dei costi della politica ha assunto particolare centralità, questa disposizione evidenzia e dimostra una chiara inversione di tendenza e un'attenzione particolare al controllo della spesa pubblica, finalizzata ad evitare sprechi di risorse già particolarmente esigue. Ma sicuramente l'ambito che necessita maggior attenzione è rappresentato dal mondo del lavoro e dalle misure necessarie per il rilancio dell'economia nazionale. In questo senso, desidero sottolineare ancora una volta, come già fatto dal presidente Sacconi, relatore per l'11a Commissione, e da altri colleghi nel corso del dibattito dinanzi alle Commissioni riunite ed in Aula, che il contenuto delle disposizioni dell'articolo 4 sugli ammortizzatori sociali in deroga può rappresentare, in questo contesto contesto di straordinarietà dovuto alla emergenza economico-finanziaria, una prima utile soluzione rispetto a questioni che stanno a cuore ai cittadini e produrre una vera boccata d'ossigeno per l'intero tessuto sociale e produttivo del Paese. Sono certamente consapevole, come pure già efficacemente sottolineato dal presidente Sacconi, che si tratta di misure di carattere temporaneo; al contempo, sono altresì convinto che il Governo riuscirà anche a trasformare le attuali politiche passive del lavoro in politiche attive, in grado di rimettere in gioco le potenzialità delle nostre imprese. Voglio a questo proposito ricordare che nel 2008 il decreto-legge n. 185, adottato dal Governo Berlusconi, ha introdotto misure a sostegno della famiglia, del lavoro, dell'occupazione e dell'impresa, ridisegnando in funzione anticrisi l'intero quadro delle politiche del lavoro. La disciplina normativa estendeva la concessione dei benefici degli ammortizzatori sociali in deroga a tutte le imprese che non potevano ricorrere agli strumenti ordinari, perché escluse da questa tutela, o perché avevano già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie. L'erogazione di queste misure era collegata alla fruizione da parte dei lavoratori di percorsi di politica attiva del lavoro, che dovevano essere programmati e attuati dalle Regioni e dalle Province autonome. L'intento era quello di preservare la base produttiva nazionale e mantenere, ovunque possibile, la costanza del rapporto di lavoro. La riforma del lavoro del ministro Fornero (legge n. 92 del 2012) ha introdotto poi novità e modifiche al regime degli ammortizzatori sociali: per le prestazioni in deroga, al fine di garantire le graduale transizione verso il nuovo regime (ASPI e mini ASPI), è stato previsto un sistema di finanziamento annuale decrescente. La riforma, confermando la disciplina della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nonché il finanziamento di quella in deroga fino al 2016, ha altresì introdotto la cornice giuridica per l'istituzione dei fondi di solidarietà settoriali cui demandare la gestione delle integrazioni salariali nei settori non raggiunti dalla cassa integrazione guadagni. In questa sede, mi limito a rilevare come negli ultimi anni si sia registrato un progressivo aumento del peso finanziario dello strumento della mobilità in deroga, che è passato dal 16,6 per cento del 2009 al 29,6 per cento La crescita della spesa complessiva per strumenti in deroga nel 2012 ha raggiunto quota 700 milioni. Ciò è dovuto anche al prolungamento della crisi, che ha ridotto le possibilità di reimpiego e di ripresa produttiva per molte aziende; al contempo, la crescita di alcune voci di spesa è da attribuire all'assenza di criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga, nonché agli scarsi strumenti di controllo delle assegnazioni regionali. In tale situazione è sorta la necessità di prevedere un immediato rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2013, così come è previsto dal decreto al nostro esame, e di far fronte all'attuale emergenza occupazionale, ricorrendo ai contratti di solidarietà e ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali. La possibilità di una proroga di alcuni contratti di lavoro a tempo determinato interessa numerosissimi lavoratori: i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato in essere al 30 novembre 2012; il personale educativo e scolastico operante negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali; i dipendenti operanti presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture - Uffici territoriali del Governo e presso gli Uffici immigrazione delle questure. Quest'ultima norma, in particolare, è intesa a garantire l'operatività sia degli Sportelli unici per l'immigrazione, in relazione ai compiti di accoglienza ed integrazione, sia degli Uffici immigrazione delle questure, per le esigenze di rafforzamento delle attività di contrasto all'immigrazione clandestina. Onorevoli colleghi, questo decreto-legge costituisce dunque la premessa fondamentale per una serie di interventi legislativi che possano creare quello *shock* finanziario che tutti auspichiamo e al quale tutti annettiamo la capacità di determinare un'inversione di tendenza. Le scelte operate con questo decreto sono senz'altro coraggiose e permettono, dopo le rigidità di bilancio del Governo precedente, di alleggerire il peso del fisco su famiglie ed imprese e di sostenere l'occupazione. Il Popolo della Libertà è infatti convinto che solo la crescita e lo sviluppo, coniugate con una diminuzione selettiva della spesa pubblica, potranno salvaguardarci da un declino che in passato è sembrato irreversibile. Per questi motivi, il Gruppo del Popolo della Libertà voterà convintamente il provvedimento al nostro esame. Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Democratico voterà convintamente a favore della conversione in legge di questo provvedimento. un ringraziamento particolare e non formale ai due Presidenti relatori - Mauro Maria Marino e Maurizio Sacconi - e ai colleghi della Commissione finanze e della Commissione lavoro per l'attento esame del provvedimento, nonostante, come è già stato ricordato, il pressante invito del Governo a rispettare i tempi per la conversione abbia oggettivamente limitato la possibilità di intervento del Senato. In questo quadro di costruttiva collaborazione con l'Esecutivo, il Gruppo del Partito Democratico non ha presentato emendamenti al testo approvato alla Camera: emendamenti che sono stati sostituiti da numerosi ordini del giorno approvati in Commissione, i quali hanno posto l'accento su diverse problematiche rilevanti, che dovranno essere affrontate e risolte, per quanto possibile, in prossimi provvedimenti legislativi e regolamentari. Di questo hanno parlato in discussione generale i colleghi Angioni, Fabbri e Moscardelli. Questo decreto-legge - giova ricordarlo in questa sede - è stato il primo atto del Governo Letta. Abbiamo apprezzato che l'Esecutivo abbia deciso di partire dall'emergenza lavoro, in particolare con il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga e dei contratti di solidarietà, nonché con la proroga della validità al 31 dicembre 2013 dei contratti dei precari della pubblica amministrazione. Lo sforzo compiuto nell'incrementare da uno a due miliardi complessivamente il Fondo per la cassa integrazione guadagni in deroga è stato significativo e ha consentito di dare una risposta reale ai problemi di reddito di decine di migliaia di famiglie e di lavoratori di aziende in crisi. L'intensità e la profondità della crisi economica e occupazionale che stiamo vivendo deve imporre al Governo e al Parlamento un'azione di costante monitoraggio del fenomeno, perché occorrerà a breve ricercare nuove risorse per rispondere alla domanda che proviene dai territori, così come è stato segnalato nelle audizioni dalle Regioni. È infatti in gioco la coesione sociale dell'Italia e, con essa, la tenuta del sistema economico e produttivo del nostro Paese. Ogni sforzo e ogni intelligenza devono essere prioritariamente indirizzate alla creazione di lavoro, alla difesa e al sostegno del settore manifatturiero, provato da una congiuntura negativa che ha caratteri e durata sconosciuti. Così come ci ha ricordato la Banca d'Italia in una recente audizione in Senato, il numero di persone in cerca di occupazione, superiore a tre milioni, ha continuato a crescere dall'inizio dell'anno. Altri 1,6 milioni di persone sono classificate dall'ISTAT come lavoratori scoraggiati, ovvero individui che dichiarano di non aver cercato un impiego perché convinti di non trovarlo. Si potrebbe continuare a lungo a snocciolare dati negativi e preoccupanti sia sul fronte della produzione che su quello dell'occupazione. Per queste ragioni riteniamo profondamente demagogico affrontare la questione dell'IMU nei termini che abbiamo ascoltato anche nelle ultime settimane. Noi lo diciamo forte e chiaro: non siamo disponibili ad avallare una strategia politico-mediatica che trasformi l'IMU in una bandiera tanto ideologica quanto inutilmente strumentale, tentando di far passare nell'opinione pubblica l'idea che questa tassa sia all'origine di tutti i mali del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Gli indecorosi e ingenerosi recenti attacchi al ministro Saccomanni rispondono a questa logica distorta e distorcente; da questi attacchi il Partito Democratico si dissocia, riconfermando piena fiducia nell'operato del Ministro. Si finisca una volta per tutte di trasmettere agli italiani una visione deformata della realtà, distogliendo l'attenzione dalle vere questioni da affrontare: lavoro e crescita. Ancora una volta richiamo l'attenzione dei colleghi su quanto affermato dalla Banca d'Italia nella recente audizione riguardante l'indagine sulla tassazione degli immobili: «L'analisi del gettito delle imposte sugli immobili mostra come l'introduzione dell'IMU nel 2012 abbia portato il prelievo italiano complessivo sulla proprietà e sugli occupanti su un livello in linea con quelli registrati nei principali Paesi dell'Unione europea». Secondo i dati della Commissione europea, nel 2011 le imposte sulla proprietà, immobiliare e non, sono state pari negli altri Paesi della UE al 2,1 del prodotto (media ponderata sulla base del PIL); le imposte ricorrenti sulla proprietà immobiliare sono state pari all'1,4 del PIL contro lo 0,7 dell'Italia. Nel 2012, considerando il gettito dell'IMU, tale ultimo valore si attesterebbe intorno all'1,5. La realtà, quindi, è ben differente dalla propaganda e la materia della tassazione degli immobili è assai più complessa di uno *slogan* elettorale da riprodurre su un manifesto per poi ripeterlo come un mantra. Grazie al meritorio lavoro compiuto dalla 6° Commissione del Senato con l'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili, oggi il Governo e il Parlamento hanno a disposizione una mappatura attenta di questa complessa materia, con una panoramica importante sulla legislazione in vigore nelle altre Nazioni europee. Bene dunque ha fatto il Governo, con questo provvedimento, a sospendere il pagamento della prima rata 2013 dell'IMU per avere il tempo di provare ad affrontare in maniera organica la questione della fiscalità immobiliare. È del tutto evidente, infatti, che la sola sospensione non può essere la soluzione finale. L'indirizzo e l'invito che oggi il Partito democratico rivolge al Governo è quello di agire secondo principi di equità e di solidarietà sociale. Per noi rimane valido quanto sostenuto in questi anni di crisi: per uscire da questa crisi è indispensabile che chi ha di più dia di più. L'esatto contrario di un'abolizione indiscriminata dell'IMU su tutte le abitazioni principali. Come dimostrano tutti gli studi indipendenti, è invece possibile agire nell'immediato con lo strumento dell'aumento delle detrazione, e ricordo che questa era stata l'impostazione inascoltata del Partito democratico Passando, ad esempio, dagli attuali 200 euro a 600 euro di esenzione resterebbero esclusi dal pagamento dell'IMU circa l'85 per cento dei

Inoltre, non può continuare a essere tassato allo stesso modo l'immobile produttivo, unico strumento della piccola azienda artigianale e commerciale, e quello costruito a scopo meramente speculativo. L'attenzione e il sostegno vero al nostro molecolare sistema di piccole e piccolissime imprese può e deve partire da qui, da una modifica del prelievo IMU sui fabbricati strumentali delle imprese artigianali, commerciali e agricole. Accanto a questi interventi realizzabili nell'immediato appare evidente come la chiave per rendere più corretto e più equo il prelievo sugli immobili passi, inderogabilmente, dalla riforma del catasto, che oggi svolge il negativo ruolo di amplificare le ingiustizie sulla tassazione, ancora una volta andando a privilegiare i patrimoni immobiliari con maggior valore di mercato cui non corrispondono corretti valori catastali. Non è credibile, infatti, che gli immobili ritenuti di lusso in Italia siano oggi solamente 73.382. Questo vuol dire che, in media, visto che le ville sono 34.628, in ogni Comune ci sarebbero quattro ville. Il catasto fotografa un'altra Italia da quella che vediamo e viviamo ogni giorno. Nell'attesa di una riforma complessiva del catasto (secondo l'Agenzia delle entrate sarebbero necessari cinque anni) potrebbero essere studiati - ed è un suggerimento che diamo al Governo - interventi correttivi per migliorare l'equità del prelievo a parità di gettito, utilizzando ad esempio nelle grandi città i dati resi disponibili dall'Osservatorio del mercato immobiliare. Inoltre - e mi avvio alla conclusione - riteniamo indispensabile che il Governo dia in tempi brevi certezza agli enti locali per quella che è diventata una delle principali fonti fonti di entrata, in ragione della progressiva riduzione dei trasferimenti statali, ponendosi l'obiettivo che l'IMU torni ad essere quella che avrebbe dovuto: un'imposta municipale unica che rimane integralmente ai Comuni. In definitiva, l'invito al Governo è quello di non cedere alle facili tentazioni demagogiche, affrontando con spirito di equità e di solidarietà sociale la modifica della tassazione sugli immobili, e parlando agli italiani un linguaggio di verità e di onestà intellettuale. Sul fronte del lavoro, o meglio del lavoro che manca, l'invito è a proseguire con determinazione il percorso avviato in sede europea dal presidente Letta; questa è la questione delle questioni non soltanto in termini economici, ma più in generale rispetto ai rischi che corre la democrazia in periodi come quelli che stiamo vivendo. Se seguirà questa strada, non facile ma necessaria per il futuro dell'Italia, il Governo avrà il nostro sostegno costruttivo e leale.

Presidente, colleghi, prendo la parola per evidenziare il grave scempio ambientale che si attuerebbe ai danni dei cittadini abruzzesi, qualora la società Snam Rete Gas realizzasse il metanodotto Sulmona-Foligno, un tubo di 167

Pizzoli, Barete, Cagnano, Montereale, Barisciano, San Demetrio, San Pio delle Camere, Fagnano e Sulmona. Stiamo parlando di un'area del Paese caratterizzata dalla presenza di faglie ad alto rischio sismico, fattore che fa inevitabilmente ed esponenzialmente aumentare i rischi in caso di realizzazione del metanodotto. In questi quattro anni la costruzione di quest'opera è stata ostacolata con determinazione dai comitati di cittadini e dalle associazioni, in quanto attraverserebbe il Parco nazionale del Gran Sasso e i monti della Laga, oltre a cinque zone a protezione speciale e di interesse comunitario.

in fatto di competenze regionali sulla localizzazione e realizzazione di gasdotti nelle zone sismiche. Il giorno 10 luglio, accogliendo il ricorso presentato dal Governo, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità di questa legge, richiamandosi alla natura concorrente della potestà legislativa sulla materia. È il caso di ricordare però che il deposito sotterraneo di gas di Rivara, in provincia di Modena, è stato cancellato dal Governo nazionale dopo che la Regione Emilia-Romagna, in base al principio di precauzione e non ad una norma regionale, ha negato l'intesa un mese prima del sisma. Quattro anni di battaglie dei cittadini e delle amministrazioni locali abruzzesi rischiano ora di andare perdute, nonostante siano in gioco valori fondamentali per la vita della nostra comunità, come il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza; eppure la tutela ambientale e del territorio dovrebbe rappresentare una delle priorità

gli esperti che si sono schierati e si schierano contro la realizzazione di quest'opera, per ascoltare e comprendere le motivazioni del

angoscia un paese, anzi direi una vallata, oltre che una famiglia. Il caso riguarda un siriano che ha ottenuto asilo politico e i suoi atteggiamenti nei confronti di una minorenne che vive in una località della Valsugana. Il ragazzo importuna sistematicamente questa minore, ottiene una condanna, il giudice ne ordina l'allontanamento da quella zona, ma il ragazzo persiste e ritorna nel paese.

Ottiene una prima condanna a otto mesi per questo atteggiamento persecutorio. Il comportamento viene reiterato; ottiene una seconda condanna; finisce di nuovo in carcere per altri tre mesi; ottiene infine un terzo arresto Per questa famiglia, non occorre dirlo, è un autentico incubo. viene sorpreso nascosto nel giardino della ragazza con l'intento di spiarla. I carabinieri, interpellati, dicono che non ci sono i presupposti per un arresto. Il ragazzo continua a dire (è la sua minaccia): Me lo suggerisce il mio Dio, la devo portare in Siria per sposarla». Vengono recapitate a mano lettere in serie

Istanbul, violenza sulle donne. Il caso non si sta risolvendo. Serve un interessamento forte del Governo, che deve assumere tutte le iniziative del caso. Dobbiamo ridare serenità a questa famiglia e sicurezza a questa ragazza, ma anche a tutta la Valle, che aspetta si faccia sicurezza e una presenza effettiva dello Stato. oggi sui giornali l'ennesima tragedia, che ha colpito - cosa orribile - due bambini, Andrea e Davide. Nonostante la madre abbia denunciato dieci volte il padre per minacce e violenze, è stata addirittura costretta a porre una telecamera sul citofono, perché probabilmente doveva ancora e ancora provare che quest'uomo minacciava la sicurezza non solo sua, ma anche dei figli. Mi chiedo cosa stiamo aspettando per agire. In questa Camera, nelle Commissioni giustizia e affari costituzionali, è in corso la discussione del disegno di legge sul femminicidio, che prevede norme molto precise per le aggravanti di violenza assistita da minore, ma soprattutto per dare la precedenza ai processi di cui

allora a tutte le donne presenti in questa Camera e in tutto il Parlamento, ma soprattutto alle donne che stanno fuori, l'invito a far sentire la nostra vicinanza a questa madre che ha gridato e non è stata ascoltata. C'è un'altra cosa che voglio denunciare. Un quotidiano nazionale, nel narrare questa tragedia, questo orrendo delitto, ha usato un tono francamente di insopportabile giustificazionismo, come se il dolore di un padre per la separazione, per l'abbandono della propria moglie propria moglie possa giustificare un così orrendo reato. Ecco, questa legge deve fare anche cultura. Per questo serve una grande mobilitazione, certo anche degli uomini, ma soprattutto di noi donne. Il mio invito alle senatrici è di andare tutte insieme, ogni volta che si riuniscono le Commissioni giustizia e affari costituzionali, ad assistere al dibattito, perché le nostre orecchie debbono sentire e soprattutto dobbiamo vigilare

a me spiace parlare quando le persone non sono presenti,

il Collegio dei senatori Questori non ha firmato alcuna autorizzazione di spesa per l'acquisto dei tesserini di riconoscimento, in quanto tale operazione rientra nelle spese autonome dell'economato. contrario, in riferimento agli inutili sprechi, ho molto da dire e ci sarebbe anche tanto da fare. È vero, l'Amministrazione poteva risparmiare circa 3.000 euro e consegnare i tesserini senza custodia, mi sembra inutile attaccarsi ai 3.000 euro, quando si potevano risparmiare 13 miliardi di euro cancellando definitivamente il progetto F-35. Ma il suo Governo non era d'accordo. caso, se vogliamo fare economie, ancora si possono fare, risparmiando circa 16 milioni di euro. Rinunciate ai rimborsi elettorali. Ora direte che non è possibile, ma non è vero. Basta non comunicare il codice IBAN e il versamento dei rimborsi elettorali non verrà effettuato. Nel frattempo potete chiedere al vostro Governo un provvedimento d'urgenza per abolirli - tanto ne fa moltissimi - e, se proprio non volete rinunciare a quei soldi, prendete esempio: noi del Movimento 5 Stelle, in circa tre mesi, abbiamo restituito un milione e mezzo ai cittadini, rinunciando ad una parte della nostra indennità parlamentare e restituendo la parte di diaria e diaria e di rimborsi forfetari non spesa. Non parlateci di sprechi quando da quattro mesi vi chiediamo di razionalizzare le spese e di impiegare le poche risorse a disposizione per salvare l'economia italiana e i cittadini italiani.